Ad un certo punto della lettura effettuata dal senatore segretario, si fa riferimento ad un intervento del senatore Caruso sull'articolo 93, in cui egli chiedeva di votare per parti separate; successivamente a quell'intervento

giusta la sintesi del processo verbale, ma noi abbiamo il diritto e il dovere di far sapere a chi leggerà questi verbali che il Governo non risponde alle questioni poste da un senatore in Aula. In questo caso si trattava di una vicenda particolarmente poco edificante. È bene che il cittadino, lo studente, lo studioso, il giurista che esaminerà i processi verbali sia messo nella condizione di sapere che il Governo non ha risposto.

gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato». A completamento di ciò vengono prodotti i Resoconti sommario e stenografico, che rappresentano comunque atti ufficiali del Senato.

Signor Presidente, per parlare di questo decreto-legge il tono forse più giusto sarebbe quello dell'ironia, se non fosse, però, che questo provvedimento naturalmente

perché tutti gli articoli successivi all'articolo 1 sono la negazione dell'articolo 1 medesimo. L'articolo 1, infatti, si presenta come il tentativo di dare rigore alla finanza pubblica, di ridurre le spese superflue, di concentrarsi sulla riduzione dell'indebitamento netto e su quella della pressione fiscale. esattamente dall'articolo 2 comincia una pletora di erogazioni che ha rari precedenti nelle pur cospicue leggi finanziarie degli ultimi anni nella Repubblica italiana. Già questo naturalmente

la dicono tutta sul valore di queste norme, che costituiscono una complessiva manovra di spesa per tenere coesa la maggioranza politica. Soltanto una lettura delle spese che sono state introdotte nell'ordinamento da questa manovra ci condurrebbe ad affermare che abbiamo effettuato esattamente ciò che non si doveva fare. Siamo in una fase in cui, per una serie di ragioni, nazionali ed internazionali, l'economia sembra volgere al peggio, comunque ad una riduzione dei tassi di crescita. In questo contesto, in cui la riduzione della pressione fiscale e la riduzione dell'indebitamento avrebbero rappresentato misure virtuose, tendenti a fronteggiare il possibile declino dell'economia, ecco che invece si fa esattamente il contrario.

Se il loro rigore è affidato allo striminzito dettato dell'articolo 1 di questo decreto‑legge, allora è davvero ben poca cosa. La verità è che questo Governo della spesa facile trova in tutti gli altri articoli di questo provvedimento solido radicamento. L'aspetto più rilevante, signor Presidente, è che ciò che aumenta è la spesa in conto corrente; questo è il punto. È vero, ci sono anche trasferimenti in conto capitale a grandi strutture

che vi sono interi settori della maggioranza che solo al pensiero della costruzione di nuove infrastrutture vitali per lo sviluppo italiano urlano improvvisamente, occupano strade, fermano treni; quindi, questa spesa si rivelerà inefficace. Peraltro, è proprio di questi giorni notizia che un Ministro della Repubblica, anzi, il ministro delle infrastrutture Di Pietro, blocca i trasferimenti a Rete ferroviaria italiana. Questo rende palese rende palese quanto sto dicendo, cioè che mentre tutto ciò che è vizioso per la spesa pubblica viene introdotto nell'ordinamento e trova il più ampio consenso di questa maggioranza, le uniche spese che forse sarebbero necessarie trovano contraddizioni non solo nei Gruppi della sinistra radicale di questa maggioranza, ma ora anche nel titolare del Ministero delle infrastrutture, colui, cioè, che dovrebbe dare impulso alla spesa in conto capitale per il rinnovamento delle infrastrutture. Un Governo, in sostanza, che si morde la coda in continuazione e non può prendere di petto i problemi che lo sviluppo dell'Italia ha di fronte, perché non ne è capace per cultura, non ne è capace per le contraddizioni politiche che la attraversano.

quasi ogni articolo di questo decreto modifica un comma della scorsa finanziaria, e lo stesso fa la legge finanziaria che abbiamo discusso in Senato. in Senato. Anche questo è il segno delle contraddizioni in cui si dibatte la maggioranza, una norma non riesce a compiere un anno di vita perché le *lobbies*, i Gruppi,

appena una norma sta per entrare in vigore, sta per esplicare i suoi effetti, ecco che qualcuno che ne è colpito porta sul tavolo della maggioranza le sue esigenze ed in tal modo le esigenze di piccoli partiti o di piccoli strati della cittadinanza italiana hanno il sopravvento sulla grande maggioranza dell'Italia che ha bisogno - ribadisco - di sviluppo e delle infrastrutture materiali ed immateriali necessarie per lo sviluppo stesso. Mancano ancora, in questo testo, norme che seriamente si pongano il problema della ricerca, cioè della conduzione del sistema produttivo italiano verso le fasce alte dei processi e dei prodotti, e dei prodotti, perché anche in questo caso i contributi per la ricerca si polverizzano in migliaia di iniziative all'interno delle quali è difficile intravedere il filo conduttore della politica governativa in questo Noi auspichiamo che istituti di ricerca possano fiorire in Italia, ma niente di tutto questo si può intravedere nel complesso normativo del quale stiamo discutendo. Non credo insomma, signor Presidente, che queste leggi servano al Paese, anzi sono profondamente convinto che continuino una delle operazioni delle operazioni economiche peggiori possibili, quella prociclica. In sostanza, si usa la finanza pubblica non per contrastare le tendenza al peggioramento dell'economia, ma anzi lo si fa sempre in maniera prociclica, cioè aumentando le tendenze negative dell'economia. Questo ovviamente non va bene per il sistema produttivo italiano. Per questo, convintamente, proporremo

più di aggiustamento delle coperture che non di carattere sostanziale e quindi vale naturalmente, quello che abbiamo detto nel corso della prima lettura al Senato. Il mio intervento molto brevemente cercherà dunque semplicemente di sintetizzare le questioni

molto importante per l'ammontare delle risorse che mobilita e per le modalità e per le destinazioni che assegna a tali risorse. Non sono d'accordo con quello che ha detto il collega Azzollini, a dire che ci troviamo in presenza di un decreto-legge interamente collocato sul versante della spesa corrente. Ricordo che 3 miliardi e 800 milioni di euro sono destinati a spese di investimento per opere pubbliche, trasporti, edilizia residenziale e ambiente

un miliardo e 950 milioni vengono destinati a spese correnti, molte delle quale indispensabili.

inoltre, pone in essere una seconda operazione, che molti colleghi hanno richiamato: individua una strategia di sostegno per i redditi bassi. Circa 2 miliardi di euro, infatti, sono destinati al cosiddetto *bonus* per gli incapienti. Si è fatta molta ironia sulla dimensione di questo intervento; si è parlato di briciole, di elemosina. Coloro che sostengono questa tesi hanno torto per due ragioni:

uno dei problemi maggiori dell'economia del nostro Paese - vi invito a dare un'occhiata ad un interessante intervento del Governatore della Banca d'Italia, dal titolo «Consumo e crescita in Italia», in cui si affronta il problema del rapporto tra crescita dell'economia, sviluppo economico ed andamento dei redditi ma anche per la natura di questo intervento che, voglio ricordarlo ai colleghi, è contabilizzato come minore entrata, riduce la pressione fiscale e compensa una fetta di contribuenti di mancati vantaggi fiscali

evidenza delle priorità e opera delle scelte a favore delle esigenze di sviluppo strutturale del Paese. C'è poi un secondo piano su cui va formulato il giudizio, ed è il rapporto tra il decreto-legge e la manovra economica.

fin dal DPEF, una scansione temporale più lenta nel percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio per tener conto delle condizioni reali dello sviluppo del Paese.

vorrei iniziare da un'affermazione del senatore Azzollini, che ha posto il problema di un giudizio ironico sul sul complesso del provvedimento perché vi sarebbe una palese contraddizione fra quanto affermato nell'articolo 1, impostato sul rigore finanziario, e quanto disposto dagli articoli successivi,

Vorrei solo ricordare che questo provvedimento, come altri del Governo sostenuti dalla maggioranza,

Il perché è presto detto: vi è la necessità di un rispetto formale delle regole dell'articolo 81 della Costituzione circa le coperture finanziarie, l'adeguatezza, la congruità e la correttezza delle risorse destinate a finanziare le norme. oggetto della discussione e sottoposto alla nostra valutazione anche un ragionamento di carattere politico, in particolare svolto dai senatori dell'opposizione: ma come - si dice - con questo provvedimento si riduce, nel passaggio tra la Camera e il Senato, il *bonus* a favore degli incapienti e poi, con la legge finanziaria, si destina al sistema delle imprese più di un miliardo di euro. Sarebbe troppo facile per me rispondere che questo è il solito giochino della destra che si colloca più a sinistra dell'ultrasinistra!

Presidente, è che la modifica era ed è necessaria per garantire agli stessi destinatari della norma, cioè i soggetti sociali più deboli, gli incapienti, di poter veramente accedere a quel beneficio ed avere veramente quei soldi entro dicembre perchè la copertura,

viene meno, secondo il ragionamento dell'opposizione, il controllo annuale sia sul 2007, perché si può andare oltre, sia sul 2008, perché bisogna rientrare. A me questa pare un'interpretazione forzata perchè la norma riguarda solo alcune Regioni che hanno intrapreso iniziative cofinanziate con l'Unione europea per finanziare appunto spese in conto capitale per investimenti. Allora non tutte le Regioni sono interessate da queste disposizioni e a me questo sembra già un elemento tranquillizzante, poi nel 2008 c'è il vincolo di rientrare.

al 2,4 per cento e credo che raggiungeremo quell'obiettivo. È vero che in queste settimane, come è stato sostenuto da più parti, anche nell'ultimo intervento del senatore Azzollini, è cambiato il quadro macroeconomico a livello generale:

dovuta alla crisi dei mutui *subprime*. Inoltre, il quadro è cambiato rispetto alla crescita europea, che è più bassa rispetto alle previsioni;

voglio ricordare che le materie prime le paghiamo in dollari e ciò avvantaggia il nostro Paese, almeno sotto questo aspetto. Certo c'è il rischio che la crescita del prossimo anno sia più bassa e quindi la possibilità di sfondamento nel rapporto *deficit*-PIL.

di garantire i settori sociali più deboli ha la possibilità, attraverso l'aumento dei consumi, di assicurare livelli di crescita adeguati per il nostro Paese. Un'ultima considerazione, signor Presidente, è d'obbligo, è stato riproposto il problema dell'aumento della spesa corrente. Desidero ricordare sommessamente che l'incremento più rilevante si è verificato nella passata legislatura, ma in ogni caso non voglio sottrarmi alla discussione.

nella passata legislatura, invece, si è finanziato l'aumento della spesa corrente attraverso l'uso dell'avanzo primario, quindi sfondando i conti pubblici e facendo crescere il debito.

Alla Camera sono state apportate poche modifiche, soprattutto miranti a garantire una copertura certa ad alcune norme di notevole rilevanza economica e sociale. Il problema delle coperture relativamente ad alcune norme, quelle più specificatamente di carattere sociale, aveva del resto suscitato perplessità anche in quest'Aula. questo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, su specifica proposta del Governo, assicurano il rispetto dell'obbligo previsto al quarto comma dell'articolo 81 della nostra Costituzione. Ciò riguarda, innanzitutto, l'articolo 44 del decreto, quello relativo al *bonus* per i cittadini incapienti. A tal proposito, mi corre l'obbligo di sottolineare che il Governo, in coerenza con il proprio programma, oltre al risanamento dei conti pubblici e agli interventi di sostegno alla crescita economica, mette al centro delle proprie scelte l'equità sociale. Purtroppo non sempre le risorse disponibili consentono di proporre misure adeguate: sicuramente non lo è l'importo di 150 euro a persona, ma è un segnale di attenzione e, comunque, è meglio di niente. Il Governo, a questo proposito, intende affrontare la materia dell'imposta negativa in maniera organica e strutturale e, in quella sede, ci si augura di poter definire importi maggiori. Lo stesso problema di copertura è stato risolto per quanto riguarda le norme relative ai soggetti danneggiati da sangue o emoderivati infetti. In sede di prima lettura del decreto al Senato, il Governo, intervenendo sull'emendamento presentato dal senatore Marino, assunse l'impegno ad adeguare lo stanziamento nella legge finanziaria: ciò è avvenuto con uno stanziamento di ulteriori 180 milioni. La volontà del Governo è quella di avviare un piano decennale per dare soluzione ad un problema che è drammatico per le persone colpite da trasfusioni infette.

ciò comunque non inficia la portata delle disposizioni sull'uso del biodiesel, la cui diffusione potrà alleggerire la nostra bilancia energetica. Dalla Camera dei deputati è stato modificato anche l'articolo 21, prevedendo che, tra i destinatari del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, si dia priorità ai soggetti sottoposti a procedure esecutive, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito. Nel decreto è stato aggiunto l'articolo 7-*bis*, su cui si è incentrata parte del dibattito in quest'Aula. Ritengo perciò mio dovere spiegare le ragioni che hanno indotto il Governo ad inserire quest'articolo nel cosiddetto maxiemendamento presentato alla Camera. Si è inteso salvaguardare, così come pressantemente chiesto dalle Regioni, la realizzazione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea. Si prevede che per il 2007 non si applichino le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, a condizione, però, che lo scostamento sia recuperato nel 2008. Le Regioni potranno quindi ottenere il previsto finanziamento sanitario integrativo soltanto se, nel prossimo anno, rientreranno dallo scostamento verificatosi nel 2007. A fine 2008, pertanto, saranno effettuate le verifiche puntuali e, se saranno positive, nel 2009 potrà essere erogato il finanziamento suddetto. Trattasi, quindi, di una norma che dovrebbe stimolare comportamenti virtuosi, tali da ottenere nelle Regioni interessate il rientro dallo scostamento conseguito nel 2007. Va sottolineato, comunque, che la norma interviene ad esercizio quasi chiuso e perciò è scarsamente incidente sui pagamenti da effettuare entro la fine dell'anno. Il Patto di stabilità, cui si è fatto riferimento, non è a rischio, per le ragioni addotte poco fa dal relatore e anche perché, oggettivamente, la norma riguarda pochissime Regioni che stanno già procedendo a rispettare l'accordo sottoscritto con il Governo. Il decreto, come è stato evidenziato dal relatore, oltre agli interventi di equità sociale contiene norme per lo sviluppo. Il senatore Curto si chiede cosa sia l'equità sociale. Credo che a lui non sfugga il fatto che lo stanziamento di 1,9 miliardi per gli incapienti e quello di oltre 3 miliardi, deciso con il decreto-legge n. 81 del 2007 a favore dei pensionati al minimo, siano un atto di giustizia e di equità sociale, cioè un atto concreto di avvio di redistribuzione delle risorse dello Stato. Si potrà dire che è poco, ma ricordo che in passato agli incapienti non si è mai dato nulla. Il significativo finanziamento destinato all'ANAS, alle Ferrovie, all'edilizia pubblica e al completamento delle reti metropolitane nelle città di Milano, Roma e Napoli, a mio avviso, è un intervento di sostegno allo sviluppo. Le infrastrutture, infatti, insieme alla logistica sono indispensabili per il sistema economico e territoriale e per attrarre investimenti. Lo sviluppo si ha non soltanto con la detassazione, come qui è stato ricordato, anche se il Governo in merito alla detassazione ha adottato provvedimenti non irrilevanti, quali la riduzione dell'IRES e dell'IRAP, la cui applicazione sinergica comporterà

Inoltre, è stata decisa la forfetizzazione delle imposte per i lavoratori autonomi, cosiddetti marginali, e per tutte le famiglie normali sono previsti l'abbattimento dell'ICI sulla prima casa, la detrazione per chi sostiene il costo dell'affitto ed altre piccole detrazioni incluse nella finanziaria dell'anno scorso o in quella in via di approvazione. L'insieme delle varie detrazioni sicuramente allevierà il costo della vita per le famiglie. La disponibilità di maggiori risorse, anche se poche, per gli incapienti e per i pensionati servirà anche a spingere i consumi interni e, quindi, a spingere l'economia del Paese perché il crollo dei consumi, come veniva ricordato dal senatore Morgando nel suo intervento e, soprattutto, dal Governatore della Banca d'Italia, incide notevolmente sulla ripresa economica. Il senatore Franco sottolineato ieri sera la necessità di puntare sulla produttività del sistema Italia in relazione anche al particolare momento di difficoltà determinato dalla crisi dei mutui *subprime* statunitensi, dal prezzo del petrolio e, per certi versi, anche dall'euro forte, anche se sull'euro le ragioni addotte dal senatore Ripamonti mi sembrano più che condivisibili. Mi permetto, però, per quanto riguarda l'euro, di ricordare che se esso ha quasi raddoppiato il costo della vita per una famiglia normale, ciò non è dipeso dall'euro in quanto tale, ma dalla mancanza di controlli nella fase di introduzione dello stesso nel nostro Paese. In altri Paesi della Comunità europea ciò non si è verificato; questa è la verità e lo dico non per polemica verso chi aveva all'epoca responsabilità di Governo. Le considerazioni del senatore Azzollini e del senatore Eufemi sulla spesa pubblica, che non sarebbe stata tagliata, sono un po' ingenerose; certo, c'è ancora molto da fare, ma la spesa corrente è stata ridotta. Rispetto al 2006, infatti, le spese correnti hanno subito una riduzione di 5,6 miliardi di euro, al netto dell'anticipato trasferimento per 11,3 miliardi all'INPS per il pagamento di prestazioni pensionistiche. Ma il senatore Eufemi, che è attento, sa bene che il tetto alle retribuzioni dei dirigenti, la riduzione del numero dei componenti dei vari consigli di amministrazione, delle consulenze e così via, non hanno ancora sortito tutti gli effetti previsti nella finanziaria 2007 e in quella di quest'anno. Ricordo, tra l'altro, che il Governo ha tagliato i tentacoli di quella piovra che era Sviluppo Italia, che negli ultimi anni era diventata rifugio per amici e parenti, fonte di sprechi e simbolo di malgoverno; questo è un dato inoppugnabile. Quindi, la strada è tracciata, il Governo intende procedere sulla strada del rigore, ma con gradualità ed equità.

prevede che le spese sostenute per finalità di sicurezza pubblica e per il contrasto alla criminalità possano far parte di quelle che evitano l'applicazione delle sanzioni a chi è inadempiente al Patto di stabilità, come previsto dall'articolo 7-*bis*. È importantissimo, in un momento in cui la questione della sicurezza è all'ordine del giorno in ogni ente pubblico e in ogni Comune dello Stato, che

intende non applicare il comma relativo del decreto-legge alle Regioni che hanno sottoscritto con lo Stato l'accordo del 30 dicembre 2004, previsto nella legge finanziaria.

una questione continuativa nel tempo, ma che gli enti sottoposti a tale misura coercitiva abbiano invece risolto i problemi di controllo del proprio bilancio.

sanzioni, al fine di avere il controllo delle assunzioni del personale, per le Regioni che invece non vi abbiano provveduto per il 2007, il rispetto del Patto di stabilità, però in via inerente al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Ebbene, visto che quest'anno, a proposito di salubrità del bilancio pubblico, sono stati concessi contributi a fondo perduto e prestiti con rimborso trentennale (è questione della finanziaria) agli enti pubblici e alle Regioni che hanno sforato il *deficit* sul piano dei servizi sanitari per quanto riguarda riguarda gli esuberi dei costi rispetto a quanto preventivato, sarebbe forse opportuno introdurre con questo emendamento una norma

interviene su una modifica del Patto di stabilità: immagino che l'obiettivo dei proponenti sia di evitare il rischio che non ci sia più il controllo annuale sul Patto di stabilità stesso.

la possibilità di sfondamento è importante perché si tratta di due miliardi di euro, e riguarda le Regioni che hanno intrapreso iniziative cofinanziate con l'Unione Europea, quindi per gli investimenti.

7-*bis*.3 modifica il vincolo del rientro nel 2008 e prevede invece di recuperare le maggiori spese

che chiedeva di poter estendere l'intervento alle spese sostenute per finalità di sicurezza e contrasto alla criminalità, nella stessa logica avrebbe dovuto esprimere un parere favorevole al nostro emendamento 7-*bis*.3

della grande intelligenza sociale del centro-sinistra, che invece si troveranno superati nelle graduatorie da cittadini extracomunitari che beneficeranno di questi sostegni, che invece non saranno a disposizione dei cittadini italiani o dei cittadini comunitari. Ripeto, complimenti. Quando andrete nelle assemblee ricordatelo ai vostri elettori, soprattutto a quelli che dite di difendere perché c'è bisogno della casa, che dite si devono aiutare: al di là delle chiacchiere, non li difenderete affatto se rifiuterete un emendamento che specifica che i beneficiari devono essere coppie di origine comunitaria. l'emendamento 21.2 tenta di individuare uno strumento di previsione. Non occorre, infatti, essere grandi maghi per comprendere che anche nel disegno delle politiche abitative dobbiamo essere più attenti al processo di inesorabile invecchiamento della società. Penso sia oltremodo giusto che proprio il Senato sia attento alle esigenze abitative, non sole delle coppie a basso reddito, ma anche degli anziani ultrasettantenni, che magari non fanno i senatori e hanno bisogno comunque di essere aiutati nell'affrontare, nell'ultimo periodo della loro vita, una questione che rappresenta una emergenza per le persone di età "normale" o media, ma che è una vera e propria tragedia umana per le persone più anziane, certamente per gli ultrasettantenni. Ebbene, il nostro è un Senato non proprio giovanissimo e pertanto dovrebbe porsi

Senatrice Bonfrisco, con questo appello apre un conflitto d'interessi rispetto ai votanti del Senato. Invito il relatore

molti dei quali hanno contratto patologie derivanti dalla manipolazione di tali prodotti e hanno subìto gli stessi danni che oggi tentiamo di riconoscere ad una parte di questi soggetti.

già avevo avuto modo di fare nel dibattito sulla finanziaria, perché sono particolarmente favorevole a questa iniziativa della Lega,

che si è sempre dimostrato sensibile e attento alla soluzione di questa straordinaria situazione. Non abbiamo oggi il tempo, ma ricordo velocemente che questo è l'unico caso in Italia verificatosi in quelle condizioni e che il vuoto normativo non ci consente di garantire una copertura economica al rischio che molti sindaci spesso corrono nell'esercizio delle loro funzioni (cosa diversa dal rischio che corrono, pur nell'esercizio delle loro funzioni, riferito ad altre situazioni e ad altri ambienti). Voglio ricordare che quel sindaco è stato ucciso nel suo ufficio da un dipendente

venne al funerale di quel sindaco in rappresentanza del Governo. Faccio, quindi, appello non solo alla sua personale sensibilità, ma anche all'impegno morale che la presenza del Governo, rappresentato dal senatore Giaretta, Grazie,

Presidente, desidero innanzitutto aggiungere la mia firma all'emendamento 34.1. Vorrei poi ricordare ai colleghi

un galantuomo che ha pagato, sul proprio posto di lavoro e per il proprio impegno sociale, un prezzo altissimo, e così la sua famiglia.

movimento che frega coloro i quali sono in attesa dei concorsi pubblici da anni e l'aiuto agli extracomunitari, dovuto quando pagano le tasse, come diceva il relatore, è molto spesso, invece, causa di discriminazione nei confronti degli italiani residenti e che lavorano nella nostra terra. Tutto ciò comporta spese per miliardi di euro. invece siamo ad elemosinare una somma vergognosa (100.000 euro) e mi stupisco di come il senatore Polledri possa avere accettato questa elemosina, anche se capisco il senso politico della vicenda. Chiedo al Governo se vi è la possibilità, anche pensando ad un altro passaggio, di affrontare questa tematica in maniera dignitosa. Poc'anzi ho sentito il senatore Polledri, al quale mi lega una grande simpatia ed amicizia, e la senatrice Bonfrisco

Non credo che la famiglia del sindaco caduto o la famiglia del sindaco di Aci Castello, caduto anch'esso in una trincea sociale e politica,

che si portano un reciproco rispetto nelle loro differenze e nelle loro peculiarità) non accettino dallo Stato questa somma e ne devolveranno sicuramente

20: andremmo a dare 5.000 euro; immaginiamo se fossero 200 o 40: andremmo a dare 500 o 1.000 euro. È una vergogna

da siciliano che sta «in piedi» (come diceva Julius Evola, scrittore al quale mi rifaccio da sempre) «in un mondo di rovine», mi asterrò pur chiedendo di apporre la mia firma, perché è una vergogna: una famiglia colpita così duramente non può accettare un'elemosina, ma soltanto un dignitoso sostegno. Questo, credetemi, fino a quando la somma rimarrà tale ed il Governo non interverrà, non è dignitoso sostegno, ma vergognosa elemosina, pur comprendendo ed approvando lo spirito con il quale il senatore Polledri ha proposto l'emendamento. *(PD-Ulivo)*. I colleghi sanno bene il motivo per cui non è possibile approvare quest'emendamento al di là del merito: il motivo che impedisce di introdurre in questo testo delle modifiche è che non sarebbe tecnicamente possibile immaginare un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Rinnovo però, con con più energia che in passato, la richiesta al Governo di affrontare definitivamente la questione. Siamo in presenza di una categoria di servitori dello Stato - chiamiamolo così perché anche i sindaci, e in particole quelli dei piccoli Comuni,

Evidentemente, c'è una volontà da parte del Governo di non arrivare ad una soluzione.

Signor Presidente, la risposta del Governo - mi spiace dirlo a una persona amica e cara che evidentemente però sottostà ad un *diktat* del Governo

Quindi, spero che voi non facciate niente, perché al sindaco siciliano hanno già pensato la Regione siciliana

ad una delle linee-guida della politica del centro-sinistra che va sotto il nome, seguendo questo articolo, di misure rivolte agli incapienti.

gerghi che spesso nascondono realtà molto più semplici e banali da comprendere: gli incapienti sono i poveri.

a favore dei poveri. non si negano a nessuno. Non sarà un ordine del giorno, come tanti ne abbiamo visti, e modificare questo stato di cose. Nella politica espressa da questa finanziaria non ci sono misure che aiuteranno le persone ad essere meno povere. Anzi, come dirò in occasione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 47, questa finanziaria renderà le persone ancora più povere. Con l'emendamento 44.1 tentiamo di ricordare gli impegni che il Governo ha assunto e di ritornare alla quota dei 300 euro per coloro che chiamate incapienti e che, in realtà, sono i poveri di questo Paese.

e le finanze*. Il Governo, sulla base delle verifiche effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, deve affermare che sulla tabella indicata non sussisterebbero le necessarie disponibilità da utilizzare per la copertura di tale emendamento.

che amano i poveri in Africa, ma disdegnano di ragionare sulle difficoltà di vita dei poveri delle loro città. Credo quindi che sia un dovere affrontare seriamente la questione della povertà nel nostro Paese. Ho apprezzato molto - anche se me lo aspettavo dal centro-sinistra - il sostegno del centro-destra al precedente emendamento; tuttavia, devo prendere atto (perché sono qui per fare politica e non per dare pugni al cielo) che l'impegno del Governo ad affrontare nel 2008 la questione degli incapienti è un risultato. So anch'io che in questo Paese gli ordini del giorno e le medaglie da cavaliere non si negano a nessuno, ma insieme dovremo lavorare perché questo diventi un concreto impegno politico. Pertanto,

di questo Governo che non prevedeva nulla a sostegno degli incapienti. Il senatore Rossi, cioè, sostanzialmente condivide la linea di un Governo

trova però le risorse per coprire uno sconto di cinque punti dell'IRES per le banche e gli istituti di credito che hanno realizzato profitti di gran lunga superiori a quelli, ad esempio, del sistema manifatturiero. Vorrei qui ricordare che, nonostante tali profitti, le banche hanno incrementato soltanto dello 0,5 per cento gli stipendi e i salari dei loro dipendenti.

Grazie,

colleghi, ho deciso con serenità e con molta convinzione di lasciare il Parlamento e il Senato della Repubblica. Per me è stato davvero un onore sedere in quest'Aula, un onore essere stato presieduto da un presidente del Senato, il senatore Marini, uomo di grande sensibilità, equilibrio e di grande valore, aver potuto lavorare in un Gruppo, la cui presidente è la senatrice Finocchiaro, di cui ho potuto apprezzare la grande forza, umanità umanità e determinazione politica e, aggiungo, il collega Boccia, che voi conoscete tutti, che unisce all'umanità anche una capacità di vigilanza notevole e assolutamente inderogabile. Ma ho avuto anche la fortuna di conoscere questa Assemblea, tutta l'Assemblea, composta da colleghi e colleghe, ascoltando i quali ho potuto sempre imparare qualcosa, Buora).* Ricordo sempre una bellissima frase che, quando ero ragazzo, giovane militante e dirigente del Partito comunista italiano, mi diceva un grande senatore di allora che qualcuno di voi, forse i più anziani, ricorderà, cioè il senatore Paolo Bufalini, che diceva sempre: «Caro Goffredo, quando stai in un'Assemblea elettiva, cerca di non fare mai discorsi propagandistici, perché devi avere sempre l'ambizione, attraverso il dialogo e il confronto delle idee, di convincere gli altri e devi avere una predisposizione costante ad essere convinto». Credo che questa sia la forza e la bellezza delle istituzioni democratiche, ragionare cioè insieme - naturalmente ognuno dalla sua parte - e tuttavia essere predisposti ad un dialogo vero che possa reciprocamente far cambiare le proprie posizioni iniziali per il bene della Repubblica italiana. Ringrazio quindi tutta l'Assemblea. Non lascio per una ragione politica, ma per una ragione personale ed esistenziale. Credo non vi sia alcuna esemplarità in questo gesto:

Lascio soltanto perché sono stato chiamato ad un impegno politico molto rilevante nel mio Partito, un nuovo partito, che è il Partito Democratico, e, per rispetto delle istituzioni, non mi considero capace

che questa attività di carattere politico si aggiunge ad un mio impegno culturale, che è la passione della mia vita, non voglio far mancare a questo Senato quell'assiduità, quell'importanza e quella disciplina che un'Aula di questo genere richiede. Aggiungo che non riesco a fare molte cose, anche perché, come mi dice sempre il dottore, sono una persona che se ne porta appresso un'altra sopra le spalle, avendo una dimensione fisica notevole. Nella mia attività quotidiana, dovendo quindi portare un peso, che è anche una fatica proprio

l'amico Piero Larizza, una persona che credo tutti conoscano e possano aver apprezzato nel corso della sua attività sindacale. Valentino).* Voglio dire un'ultima cosa: naturalmente, lasciando il Senato, cercherò di fare tutto il possibile per rafforzare il mio Partito, per difendere e impegnarmi per la mia causa. Tuttavia, voglio dire che il mio impegno sarà anche perché il Partito Democratico possa contribuire a creare in Italia un bipolarismo più stabile, più civile, meno forzoso, dove si confrontino in maniera più omogenea diverse ipotesi politiche e diversi schieramenti, più coerenti, più omogenei e meno

con questo piccolo finale di buoni propositi politici, buon lavoro e vi ringrazio se potrete accogliere le mie dimissioni già da subito al primo voto, perché credo che, dopo un discorso così semplice e sincero, non vi sia bisogno di fare gesti di buona educazione formale.

il modo con cui il collega Bettini chiede di approvare le dimissioni, induce il Gruppo di Alleanza Nazionale a votare a favore. Non è vero, senatore Bettini, che lei non faccia questa mattina un gesto esemplare: chiamato ad occuparsi del partito, rinuncia a fare il senatore. Avremmo gradito che anche altri, chiamati a dirigere il partito, avessero fatto lo stesso suo gesto, rassegnando le dimissioni da sindaco della città di Roma.

perché negli ultimi anni si è arrivati alla politica da altre strade, ma ci sono quelli (come noi e come lei, senatore Bettini) che, su fronti diversi, hanno leccato francobolli, hanno attaccato manifesti e considerano il partito lo strumento che ci consente di fare tutto quello che facciamo: il partito diventa quindi la cosa più importante,

Grazie, senatore Bettini.

ma ho la sensazione che, dopo il discorso del senatore Matteoli, le dimissioni saranno accettate e quindi, a differenza sua, io terrò sospeso il buon lavoro o no, perché i cambiamenti di questi giorni non mi fanno intuire se Bettini sarà un avversario o un alleato: per questo non gli dico buon lavoro, ma nemmeno il contrario. Per onestà intellettuale, però, senatore Bettini, pur essendo il voto segreto, senza impegnare il Gruppo nel quale ho l'onore di militare, con molta onestà, dichiaro che voterò contro, per una ragione tutta politica. Noi infatti attraversiamo un dibattito sulla natura del ruolo del parlamentare,

i segni della "casta" e siamo gente semplice che sta tra la gente ma facciamo i parlamentari - una sorta di bollino, ma negativo, che noi stessi abbiamo fabbricato, cui saremmo i nominati. Persino una figura che unifica tutti noi, per la stima che ha conquistato in questi mesi, il presidente Napolitano, ci ammonisce ogni tanto che bisogna ritrovare una legge elettorale che leghi al territorio. Se mi permettete, credo che nostra prioritaria funzione sia di fare leggi, di essere legislatori, e nell'Italia del federalismo, dove la straordinaria parte delle funzioni del Governo, non già del Parlamento, è e sarà sempre di più delle Regioni, dei Comuni e degli enti intermedi, mi dà un po' la mosca al naso la pretesa che il legislatore debba avere un rapporto con il territorio come se il nostro compito fosse quello di gestire rapporti come farmacisti - con rispetto della categoria di cui ho sposato anche un membro - e non invece quello di scrivere leggi. Pertanto, colleghi senatori, già ci dicono che siamo nominati, che non rappresentiamo nessuno, che siamo i figli dei partiti, se ci mettiamo pure a dimetterci noi a seconda delle esigenze di partito, temo che il bollino ce lo rendiamo indelebile nel momento in cui invece avremmo tutti bisogno di nuotare contro la corrente della demagogia che, con il pretesto dei parlamentari nominati,

ha sfatato l'antico mito dell'assenteismo, che in questa legislatura non c'è perché credo che entriamo nel libro dei primati della Repubblica italiana come la legislatura in cui tutti i senatori hanno lavorato di più.

molta correttezza e amabilità il senatore Bettini mi ha anticipato, incrociandomi in Aula, quella che sarebbe stata la sua intenzione e le sue motivazioni, che comunque già conoscevamo per averle apprese da notizie di stampa. Non ho avuto alcuna difficoltà ad anticipargli i nostri auguri di buon lavoro, anche perché dimissioni come queste, che appartengono a scelte di etica politica, non possono, secondo noi, che essere apprezzate: di solito si lascia il Parlamento per altri motivi, non certo perché chiamati a svolgere un ruolo che parallelamente può essere coniugato anche con l'attività parlamentare. Ecco perché anticipo - come ha fatto a nome di altri colleghi del centro-destra il collega Matteoli - il nostro voto favorevole, augurandomi che l'appello del collega Castelli possa essere accolto, nel senso che, se vogliamo lavorare affinché questo Parlamento possa essere espressione di culture, intelligenze e sensibilità diverse ma sempre coniugate all'interno della logica politica, e non del vituperio, non dell'accusa pesante di carattere personale e dell'ingiuria, la politica attraverso la creazione anche di un nuovo scenario, del nuovo Partito Democratico, possa fare la propria parte allorquando sarà chiamato

di voto a favore delle dimissioni con motivazioni che riguardano anche un decennio di vita vissuta. Molti colleghi hanno ascoltato il tuo intervento, Goffredo. A me ha colpito molto - e qualche giornalista scriverà "ovviamente" - quel tuo riferimento al bipolarismo coatto. Molti non sanno dove prospera, il coatto: in quelle borgate dove c'è sofferenza, in questa città dove molto spesso si risponde all'accerchiamento che l'individuo avverte su di sé con atteggiamenti di tracotanza. Lì prospera la pianta del coatto, tutti fanno muro, qualcuno emerge come capo del branco e si circonda di tutte quelle persone che adottano quel tipo di atteggiamento. Mi sembra che questa sia la natura delle coalizioni come l'hai individuata. Io la penso diversamente, credo sia molto diverso, ma credo anche che bisogna portare profondo rispetto verso questi percorsi politici. Viviamo in una città in cui, per cinque anni, è andata bene a noi: penso alla Provincia, alla Regione, al Governo. Per cinque anni ci siamo confrontati, io alla testa di questo schieramento tu alla testa dell'altro. Nei cinque anni successivi ha vinto la sinistra ed io non potrò mai dimenticare i riconoscimenti leali che ci sono stati in questo percorso. Desidero ricordare una persona a cui abbiamo voluto bene entrambi, alla quale hai dedicato una riflessione amara, in quel momento, per il tuo partito, ma molto importante. Quando la destra vinceva in questa città dedicasti una riflessione al fratello di un nostro senatore, Antonio Augello, consigliere comunale in Campidoglio, persona che hai rispettato e che tutti hanno rispettato. Ricordo quell'episodio perché fa parte del tratto garbato di una persona dura di convinzioni, ma sicuramente capace di ascoltare. Ti raccomando solo una cosa nell'attività che intraprenderai da domani, se il Senato approverà le tue dimissioni: fai capire a tutti che l'opposizione è fatta di persone serie. Ha ragione il senatore Castelli nel dire che le tue argomentazioni dovrebbero motivarci a votare contro le dimissioni. Avremmo interesse a rendere più difficile il tuo lavoro, a costringerti a stare in Aula a votare, a dover sperare che manchi uno di noi, a far sì che la coalizione non abbia nemmeno un voto in meno e magari a farti fare male il lavoro a cui il segretario del tuo partito ti ha destinato. Ecco, noi facciamo il contrario, proprio perché rispettiamo le persone

L'altra raccomandazione che vorrei farti, visto che l'hai buttata in politica, è di dire a Veltroni che la politica non si fa soltanto con gli accordi di Palazzo perché la gente fuori non ne può più. Presidente, senatore Bettini, è ovvio che quando si presentano dimissioni il voto dei singoli senatori e deputati è totalmente libero; quindi, non parlo a nome del Gruppo UDC, perché ciascuno dei colleghi voterà come riterrà opportuno. Mi auguro che votino a favore dell'accoglimento della richiesta di dimissioni per una ragione che il collega Bettini ha avanzato, non buttandola in politica, caro amico Storace,

alcune considerazioni in ordine alla decisione prospettata dal collega Bettini di dimettersi dal Senato e alla richiesta di

Non a caso è stimato dal mondo politico in generale, proprio perché esprime una raffinatezza dell'azione politica che raramente si incontra

dovessi dire che ho sempre condiviso nel percorso di questi anni le posizioni specifiche di Goffredo Bettini direi qualcosa di non vero e quindi di non rispettoso nei suoi confronti. Certo, Goffredo Bettini ha svolto funzioni molto importanti e molto delicate nell'organizzazione di ciò che oggi è Roma, nel bene e nel male, sia da consigliere comunale, coordinatore di una maggioranza che aveva anche impostato un progetto di sviluppo, un progetto di nuova tessitura politica a Roma, sia nelle fasi in cui si è gettato con molto entusiasmo e con molta capacità nell'avventura dell'Auditorium, che porta Roma ad uno dei livelli più elevati della produzione culturale e artistica del nostro Paese, sia - immagino - adesso che viene chiamato a svolgere una funzione delicata, come sempre di cerniera, di interlocuzione, di tessitura, che fa parte delle caratteristiche proprie di Goffredo Bettini. È evidente che in questa azione di tessitura il partito di Rifondazione comunista, non soltanto a Roma e nel Lazio, ma, a livello nazionale, avrà modo di confrontarsi con molta determinazione, con molta chiarezza e, come sempre, con grande trasparenza e lealtà. e lealtà. Francamente non siamo interessati a queste declinazioni del bipolarismo, dolce, meno dolce, amaro, completamente amaro, con poco zucchero o macchiato come un cappuccino. Pensiamo di essere oggettivamente in una condizione politica di stallo, che richiede una riforma, anche elettorale, insieme a quella istituzionale. È noto che da questo punto di vista le nostre posizioni sono rivolte a recepire nell'ordinamento italiano lo schema di legge elettorale sul modello tedesco, che garantisce stabilità dei Governi ma effettiva rappresentanza e rappresentatività politica e sociale. Si tratta di un dato privilegiato da parte nostra, anche perché l'idea che la costruzione bipolare possa contenere e contenga in effetti questi elementi di trasversalità spuria ci fa sorgere qualche qualche preoccupazione rispetto alla necessità di tirare fuori il nostro Paese dalle condizioni di ambiguità in cui oggi vive. di buon lavoro a Goffredo Bettini, da questo punto di vista, è davvero sincero. So che Goffredo è nelle condizioni di esprimere, nell'incarico che è chiamato a svolgere, una funzione importante e decisiva, ma saprà anche organizzare il confronto e l'ascolto con gli altri interlocutori. Presidente, ringrazio Goffredo Bettini per il lavoro di quest'anno e mezzo. Lo faccio tra l'altro a nome dei senatori e delle senatrici di questo Gruppo, che dall'altro ieri si chiama Gruppo del Partito Democratico-L'Ulivo. Anche il cambio di denominazione di questo Gruppo, con quello che significa, è frutto del lavoro di Goffredo, a cui auguriamo di continuare bene, con serenità e con la capacità che ha sempre dimostrato, il lavoro che ha appena intrapreso. Vorrei associarmi ai colleghi che nell'occasione di questa richiesta di dimissioni hanno dato atto a Goffredo Bettini di aver saputo interpretare nel nome e nel modo in cui ci piacerebbe fosse interpretato anche da noi stessi

Credo anche che non debbano pronunciarsi i Gruppi, per ragioni istituzionali. Personalmente voterò a favore delle dimissioni. Credo che in questo caso sia giusto non seguire la prassi consueta. Naturalmente, se non avessi sentito il suo discorso avrei votato con più convinzione a favore delle sue dimissioni, perché egli ha svolto considerazioni di politica molto opinabili, sulle quali però non è questa la sede per soffermarsi.

Presidente, non capisco il significato del dissenso, poiché il voto è a scrutinio segreto e quindi non mi pare vi sia una linea di condotta da seguire. Voterò contro la richiesta di dimissioni del senatore Bettini perché mi ha convinto il suo discorso.

luce del discorso che ha fatto questa mattina, darebbe a noi tutti una bella lezione e un bell'insegnamento. Per questa ragione, come

avevo chiesto di parlare all'inizio ed ho avuto anche una trattativa con i collaboratori della Presidenza in relazione al titolo su cui avrei

la dichiarazione a titolo del Gruppo: qui ciascuno rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato in questo specifico atto di accettazione. vorrei solo dire che ho compreso perfettamente il senso del suo discorso e vorrei chiedere a lui, ma a tutti i colleghi, di fare un passo in più: egli ha deciso di lasciare il Parlamento per dedicarsi al partito, perché il partito gli ha chiesto di dedicarsi a tempo pieno al suo nuovo ruolo e lui, tra il Parlamento, cioè i cittadini che lo hanno eletto,

di negativo e nulla di scandaloso, ma voglio solo far notare al collega Bettini e agli altri colleghi che egli è stato un nome importante per la campagna elettorale campeggiava su tutti i manifesti elettorali. Quindi, in qualche misura, la sua presenza superava anche l'obiezione che viene fatta rispetto alla legge elettorale, per la quale saremmo dei nominati dei partiti. partiti. Signor Presidente, si è polemizzato contro gli eletti con questa legge elettorale e si è sostenuto che una delle ragioni per cui la legge elettorale debba cambiare è che il sistema di selezione sarebbe sbagliato e lontano dal diritto del cittadino di scegliersi i suoi rappresentanti. di quello del collega Bettini, nel quale il nome sulla lista ha trascinato il voto dei cittadini. Con le sue dimissioni egli affida totalmente al partito il suo ruolo di parlamentare.

Nell'accogliere le dimissioni del senatore Bettini, mettiamo la parola fine alla demagogia sull'elezione o sulla nomina. Non vorrei più sentir parlare, in questo contesto e in ogni altro contesto politico, questa distinzione, soprattutto adesso che ci accingiamo eventualmente a riformare la legge elettorale.

che il Senato non assecondi le richieste in base a chi viene eletto segretario di partito.

Colleghi, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Bettini. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto. I senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra. I senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

Al senatore Goffredo Maria Bettini rivolgo, a nome dei colleghi, un cordiale saluto. Per consentire alla Giunta delle elezioni di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore dimissionario,

La seduta è ripresa. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre

ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista a cui apparteneva il predetto senatore è Pietro Larizza. Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Pietro Larizza. *(Applausi).* Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

notevolmente infastidito dall'editoriale «Le prediche di Marini» apparso sul quotidiano "l'Unità" di oggi. Ritenevo personalmente che fosse stato detto da tutte le parti e che nulla vi fosse da aggiungere. Avevo pensato di dare al mio intervento un taglio del tutto diverso da quello che invece a partire dal fatto che avevo pensato di dar lettura sia dell'articolo che il senatore Furio Colombo ha avuto modo di pubblicare su "l'Unità" del 27 ottobre dello scorso anno sia di altro articolo reperito sulla pagina "pigrecoemme.com" di Internet, in cui si faceva riferimento agli incarichi ricevuti dal senatore Colombo. Chi vorrà, avrà modo di andare su Internet e farsene una conoscenza personale. Cambio completamente il taglio del mio intervento, Presidente. Sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni del senatore e, se mi consente, amico, Goffredo Bettini che condivido quasi integralmente. Siamo stanchi credo tutti quanti da questa e dall'altra parte dell'emiciclo di comportarci come si era usi fare quando i rossi ed i neri avevano ridotto le aule di giustizia come gli ippodromi di Bisanzio. Siamo stanchi di partecipare a uno scontro continuo, spesso assolutamente strumentale a interessi non apprezzabili e spesso, invero, assolutamente sterile. Ha ragione il senatore Bettini quando parla di un bipolarismo mite, se si vuole, e non coatto. Aggiungerei che probabilmente, mutuando anche io una frase tipicamente romana, il bipolarismo, per essere mite e non coatto, ha necessità di un altro detto romano: «volemose bene». Nella realtà, ciò non significa mettersi d'accordo, ma non volerci del male; comprendere in termini chiari che ciascuno di noi può avere idee completamente diverse da quella dell'altro in maniera legittima; che nessuno di noi è proprietario della verità e che ciascuno di noi, quando manifesta il proprio pensiero, deve essere presunto, sia pure - come si dice nel mondo del diritto - *iuris tantum,* in buona fede. fede. Cosa c'entrano, signor Presidente e onorevoli senatori, nella critica legittima che ognuno può rivolgere alle posizioni dell'altro, gli insulti di natura personale? Ieri sono intervenuto per segnalare, per un verso, al Presidente del Senato cosa era stato detto sul Senato e, per altro verso, perché ero rimasto stizzito - questo sì, davvero tanto per essere stato appellato come teppista, come un uomo che non ha alcuna immagine da difendere e come il servo di un padrone. È tutto qua

io non ho mai offeso, in modo più o meno incredibile, la senatrice Levi-Montalcini, nei cui confronti va, in modo assoluto, la mia stima. Io non l'ho mai offesa e sfido chiunque a dimostrare il contrario sulla base del Resoconto stenografico di quella seduta, che riporta il mio dire considerazione, signor Presidente, è che io ho dedicato la mia vita al servizio della mia famiglia, pur nelle modifiche ha dovuto subire nel trascorrere del tempo, e al servizio dello Stato. mi dispiace davvero tanto che in questo editoriale si debba leggere di Nitto Palma (in seguito sostanzialmente definito come un bandito) la sua carriera di magistrato a Roma rifulge solo per la preziosa amicizia con Cesare Previti. Non avrei detto una sola parola se si fosse scritto che la mia esperienza umana rifulge per l'amicizia con Cesare Previti, ma non è quello che è stato scritto, quasi a voler suggerire che l'amicizia e la mia funzione di magistrato abbiano mai potuto avere delle commistioni. Siccome non ho davvero timore di nulla, sul punto sfido chiunque a dimostrare il contrario. La mia vita rifulge anche per l'amicizia nei confronti di Cesare Previti, ma la mia vita di magistrato, signor Presidente, signori senatori, rifulge - se rifulge per l'impegno che ho avuto nei processi di terrorismo, di criminalità organizzata ed è qui davvero inutile farne l'elenco perché sembrerebbe quasi un atteggiamento di vanagloria. Questo intendevo dire perché lo debbo nei confronti dell'unico valore che ho, dell'unico valore serio che posso trasmettere ai miei figli, cioè la dignità del mio nome.

Grazie,